una valutazione da parte del Governo, in sede di emanazione del decreto, rispetto al parere delle Commissioni parlamentari - naturalmente del tutto legittima - vorremmo conoscere la sua opinione sul tema dell'applicazione del massimo ribasso, ovvero sulla soglia del milione

Ne ha facoltà. MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Ministro, l'articolo 178 del nuovo codice degli appalti stabilisce che, per le concessioni autostradali che scadono entro aprile 2018, la procedura per la gara vada avviata nel più breve tempo possibile. La concessione piemontese della ATIVA scade tra soli tre mesi e la Torino-Piacenza tra un anno. Le procedure, quindi, avrebbero già dovuto essere avviate da tempo, poiché richiedono circa due anni per giungere al termine, e ogni giorno di proroga implicita determinato da questo ritardo frutta al concessionario - guarda caso, è lo stesso per le due - mezzo milione *extra* di profitti. Le chiedo allora quando verranno indette le gare per queste due tratte. Quanto all'articolo 183, le Commissioni di Senato e Camera avevano chiesto di inserire l'esclusione dell'applicazione del cosiddetto *project financing* per il rinnovo delle concessioni, perché non c'è alcun progetto nel rinnovare una concessione, a meno che non lo si usi in modo strumentale. Il fatto che il Governo abbia disatteso il parere pressoché unanime di entrambe le Commissioni vuol dire che intende applicare questo articolo? Intende applicarlo anche alle due concessioni che ho citato precedentemente, azzerando praticamente le gare, perché le altre due concessioni in scadenza sono state, di fatto, rinnovate con il metodo *in house*, usato peraltro in modo improprio? Mi riferisco alle autostrade del Brennero e alle autovie venete. Lei stesso ha più volte dichiarato che, per il rinnovo delle concessioni, la gara deve essere la regola e non l'eccezione. Per adesso abbiamo visto solo eccezioni e allora vorremmo vedere la regola almeno una volta, signor

Un particolare regime transitorio è previsto per le concessioni autostradali scadute, ovvero per le quali la scadenza viene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, al fine di procedere all'affidamento secondo procedure di evidenza pubblica. Ebbene, l'autostrada Brescia-Padova è stata affidata in concessione nel lontano 1956. La scadenza della concessione è stata varie volte prorogata e con la convenzione del 2007 sarebbe ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2026, in funzione, però, della realizzazione della Valdastico Nord, il cui progetto definitivo sarebbe dovuto, tuttavia, essere approvato entro il 30 giugno 2013, e siamo nel 2016. Il 16 maggio 2016 ha dichiarato che è stato trovato l'accordo e che la Valdastico si farà, ma non l'autostrada, bensì un corridoio infrastrutturale di interconnessione tra il Trentino e il Veneto. In questo modo, confermando la concessione dell'autostrada più trafficata d'Italia senza gara pubblica, oltre un miliardo di euro di patrimonio pubblico andrà ai privati e i pedaggi per i cittadini continueranno a essere elevatissimi. Alla luce di quanto premesso, si chiede: luogo, quali sono le motivazioni e l'opportunità politica che porterebbero a confermare la proroga della concessione dell'autostrada Brescia-Padova senza procedura di gara; in secondo in base a quale titolo la società concessionaria dal 2013 continua a esercitare la concessione dell'autostrada Brescia-Padova in mancanza di approvazione del progetto previsto definitivo della Valdastico Nord. il nuovo codice degli appalti è entrato in vigore dopo una sorta di affanno cui questo Governo ci ha ormai abituati, per rispettare scadenze senza adeguati tempi di metabolizzazione, con il concreto rischio di disorientamento e necessità di proroghe tecniche. Si tratta tuttavia di una nuova era per i lavori pubblici, caparbi e coraggiosi nell'utopia di porre fine ai tanti sistemi in calza che hanno funestato il nostro Paese. È alla luce del nuovo codice, quindi, e dei poteri conferiti all'Autorità nazionale anticorruzione, nella persona dell'attuale presidente Raffaele Cantone, che mi preme di sapere come il Governo intenderà affrontare le molteplici criticità degli appalti già in essere e in corso d'opera inerenti il settore dei trasporti, che attraverso varie interrogazioni, tutt'ora inevase, ho sottoposto all'attenzione dell'Esecutivo. Si tratta di *focus* specifici, che riguardano direttrici fondamentali per la mobilità del Paese. Ne cito alcune. E ho continuato a denunciare, come Sinistra Italiana, in sede di Commissione lavori pubblici, lo scempio della quarantennale storia di sprechi ed errori di progettazione riguardanti l'eterno cantiere della autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quadro del generale dissesto idrogeologico che rischia di affossare il Paese. E ho ribadito, alla luce dei crolli e degli incidenti mortali che si sono verificati, la necessità di misure di messa in sicurezza e soluzioni definitive per il cantiere. Non si contano più le interrogazioni che ho presentato sulla vicenda infinita dell'autostrada Tirrenica, su cui il Governo nicchia e non risponde. Il 18 febbraio 2015, durante un'audizione in Commissione lavori pubblici, proprio sulla riforma del codice degli appalti, ho chiesto al presidente Cantone di focalizzarsi su una serie di opacità. Il 10 febbraio avevo già depositato in Commissione un'interrogazione urgente per sapere con quali criteri l'allora ministro Lupi intendesse procedere nella realizzazione del progetto, alla luce della procedura di infrazione europea aperta per le irregolarità presenti nella convenzione tra ANAS e Società autostrada tirrenica. Nei mesi scorsi ho riproposto la questione, depositando una nuova interrogazione. Sulla Tirrenica, come sui crolli della Salerno-Reggio Calabria, credo credo sia necessario applicare un intervento di sistema, che metta in maniera non estemporanea a *focus* determinati eventi, spesso disastrosi.

La certezza che abbiamo sulla riforma del codice degli appalti - e siamo stati facili profeti - è che dalla sua immediata applicazione avremmo avuto sicuramente dei problemi. E i problemi li ravvisiamo non solo noi, ma anche

criticità, visto - mi permetta di dirlo - il pessimo lavoro fatto nell'altro ramo del Parlamento. Noi vogliamo ancora una volta, signor Ministro, essere propositivi verso questa riforma del codice degli appalti, perché siamo consapevoli che è importante per il nostro Paese. ragione per cui la settimana scorsa le Commissioni lavori pubblici congiunte di Camera e Senato, riunitesi alla Camera, si sono date un *timing* di lavoro, dicendo che da giugno andremo avanti con delle

BRUNI *(CoR)*. Signor Ministro, anch'io ritorno sulla questione del nuovo codice degli appalti,

è entrato in vigore senza *vacatio legis* - questo è un altro problema segnalato dal Consiglio di Stato - e presenta una serie di errori formali, con citazioni di articoli che non ci sono e che vanno corretti. A tutto ciò aggiungerei quanto è già stato detto prima l'eccessiva possibilità di fare riferimento alle gare al massimo ribasso con la soglia fino a un milione, che costituiscono l'80 cento. E, per quanto riguarda l'offerta economicamente più vantaggiosa, la partecipazione dei membri della commissione a sorte sopra i 5,2 di euro scelti nell'elenco dell'ANAC è una cosa abbastanza riduttiva. Come ultima considerazione, il *rating* di legalità riguarderebbe solo le imprese con fatturato superiore a due milioni. La domanda che

potranno essere apportati a queste criticità, che già si sono evidenziate in circa un mese di applicazione del codice degli appalti? Infine, le chiedo chiarimenti sul buco che riguarda il *rating* di legalità per le imprese sotto i due milioni

di recepimento e di attuazione più importante è in fase di avanzata predisposizione. Non ci sono vuoti, perché ogni articolo, laddove necessiti di un provvedimento attuativo, rimanda

nuovo che il massimo ribasso è molto meno pericoloso nel momento in cui va a gara un progetto esecutivo.

Noi abbiamo scritto che, sotto la soglia, le stazioni appaltanti possono scegliere dei componenti.

il momento in cui viene firmata dal Presidente della Repubblica, e non il momento in cui viene pubblicata. Ritengo un vantaggio che il Governo italiano rispetti le scadenze e un fattore di serietà. Abbiamo fatto in tempo. Quanto alle certezze e ai problemi, il senatore Crosio ci richiamava a mantenere aperto un dialogo e a tener presente il lavoro che voi farete. Certamente noi lo seguiamo con grande interesse, come abbiamo fatto anche in precedenza. È evidente che poi il Governo ha assunto

assolutamente. Il Governo è pronto ad ascoltare e recepire le vostre sollecitazioni, che sempre hanno permesso di arricchire la discussione. Per quanto riguarda il tema dei *project financing*,

La Brescia-Padova ha ottenuto un prolungamento di concessione dalla Unione europea fino al 2026. Quindi, la sua concessione non è stata prorogata, bensì è in essere fino al 2026. L'Unione europea, concedendo tale prolungamento, ha contestualmente detto che la concessione poteva essere revocata nel caso non si trovasse una soluzione alla costruzione della Valdastico. La costruzione della Valdastico, cioè del corridoio che collega la provincia di Trento al Veneto,

a costruire un corridoio che - come tutte le opere che ho intenzione di promuovere - per il quale non vi è *overdesign*. È inutile realizzare autostrade a pedaggio con sei corsie, tre per senso di marcia,

Non c'è stata quindi alcuna proroga e non abbiamo intenzione di concederne attraverso procedure strane come il *project financing* ad ATIVA o alla Torino-Piacenza. Sono già partite le procedure che istruiscono dette pratiche.

dobbiamo procedere rapidamente. Il senatore Cervellini ha sottolineato lo stato disastroso dei lavori pubblici italiani e io concordo con lui. Credo che il codice dei contratti ci consenta di compiere un notevole passo in avanti. Sappiamo che questo è un cambio di orizzonte completo.

perché sono l'elemento che darà la massima garanzia di trasparenza anche nell'applicazione del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

di avviare la procedura, anzi dice che è addirittura già avviata, e quindi la prendo in parola. Nei Parlamenti che si rispettano la parola del Ministro è molto importante per entrambe le parti e noi speriamo di essere un Parlamento che si rispetti. Per quanto riguarda gli affidamenti *in house*, su questo come su altri argomenti, può darsi che qualcosa sia concesso dall'Unione europea, ma dobbiamo innanzitutto rendere conto ai cittadini italiani più che ai burocrati europei: se una cosa conviene ai cittadini italiani, facciamola anche se i burocrati europei non la consentono. Inoltre, fare le gare secondo il codice degli appalti è conveniente, anche quando l'alternativa è darli a una partecipata molto vicina ai partiti di Governo.

A4. Nell'interesse pubblico doveva essere revocata la concessione, essendo venuta meno la condizione della costruzione dell'autostrada. In tal modo, il valore miliardario della concessione sarebbe finito nelle casse dello Stato piuttosto che nelle tasche dei privati. Signor Ministro, al danno poi si aggiunge la beffa.

Sud. Tali scarti industriali minacceranno la salute di migliaia di cittadini per anni e anni a venire. Signor Ministro, è significativa la sua risposta ed è assolutamente doveroso prenderne atto.

perché così com'è è sicuramente migliorabile. Sono contento della sua rassicurazione. Lavoreremo gomito a gomito con il Governo e la volontà di riaprire la linea di credito del Parlamento verso il Governo potrebbe funzionare potrebbe funzionare anche in virtù del fatto che questa volta Camera e Senato lavoreranno nella stessa stanza, per cui il passaggio da un ramo all'altro non ci consegnerà i problemi che abbiamo sul codice degli appalti, che sono stati generati proprio dai vari passaggi. Mi dichiaro a questo punto discretamente soddisfatto. Ci conosciamo, ma le staremo comunque con il fiato sul collo, perché apprezziamo la sua onestà intellettuale. Vorremmo, però, che tutto il Governo - ripeto, tutto il Governo - mantenesse questo atteggiamento e ci permettesse di lavorare in tal senso. Facciamo ancora un tentativo. Confidiamo in lei più che nel Primo ministro, da questo punto di vista. *(CoR)*. Signor Ministro, prendo atto delle sue risposte e segnalo che, per quanto riguarda il problema del *rating* d'impresa, andrebbe studiata meglio la situazione perché o si applicano dei criteri generali a tutte le

Voglio prendere atto ulteriormente della sua dichiarazione sull'attuazione delle opere, che è l'obiettivo del Governo. A questo proposito penso che i correttivi

recente, ossia la Maglie-Leuca, che non può essere una strada appaltata a due imprese contemporaneamente, o meglio con pronunce della magistratura amministrativa contrastanti, lasciando un territorio così importante senza un'arteria stradale di grande collegamento.

ORRU' *(PD)*. Signor Ministro, esprimo apprezzamento sullo schema di decreto legislativo recante «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994», che abbiamo appena incardinato in Commissione lavori pubblici per il parere. Questa riforma si inserisce perfettamente nel solco della stagione di riforme che il Governo sta portando avanti, rispondendo alla precisa necessità di consentire al nostro Paese, anche in tema di portualità, di cogliere le opportunità di crescita e di sviluppo che merita, contrastando la perdita di competitività che i nostri porti stanno subendo rispetto a quelli europei. Ci sarebbero, però, alcune questioni non previste nello schema ma che appaiono rilevanti. Nella fattispecie, per corrispondere nel miglior modo possibile all'architettura istituzionale delineata che vede la transizione da autorità portuale oggi prevalentemente mono scalo ad autorità di sistema portuale prevalentemente multi scalo, a nostro avviso sarebbe opportuno che i porti dei Comuni capoluogo quali Trapani, Oristano, Crotone, Vibo Valentia, Barletta, Pesaro e Pescara, attualmente non sede di autorità portuale, vedessero una propria rappresentanza all'interno del comitato di gestione, al fine di non dare la sensazione di un esproprio del porto del proprio territorio, ma al contrario per poterne beneficiare massimamente. Ovviamente è opportuno valutare e prevedere tutte le possibili implicazioni, a partire anche da un'eventuale pesatura del ruolo che il rappresentante del territorio eserciterebbe nel comitato di gestione. Al riguardo, signor Ministro, le chiedo quali sono le intenzioni e se sono attualmente allo studio misure finalizzate in merito a quanto richiesto.

guardare con attenzione ai territori, all'intermodalità, alla connessione delle merci e dei passeggeri. Tuttavia, la semplice riorganizzazione delle autorità portuali non risolve il problema del nostro Paese Paese di connettere correttamente l'ultimo miglio ferroviario con il porto o l'aeroporto, con le strade o con l'interporto, e di rendere i nostri porti

a valle di questo provvedimento fondamentale e importante - lo accelereremo per l'approvazione - il Governo mette a disposizione delle risorse economiche importanti perché poi

Come intende recepire e in quali tempi le eccezioni sollevate dal Consiglio di Stato e, in particolare, sulle gare europee per le concessioni, anziché la procedura ad evidenza pubblica che - secondo il Consiglio di Stato e come sostengo da sempre - lascia troppa discrezionalità alle autorità portuali? Cosa potrebbe accadere a tutte le proroghe di concessioni recentemente rilasciate, con disinvoltura e in modo inopportuno da alcune autorità portuali italiane anche per decenni, mentre lei peraltro stava emanando il regolamento per il riordino dei porti,

conoscere i criteri di scelte, competenze e conseguenti nomine dei presidenti delle autorità portuali e in quali tempi, anche per chiudere le sterili polemiche sulla mancanza di gestione dei porti da parte dei commissari, del tutto immeritate e strumentali, portate avanti da chi vorrebbe solo facili proroghe senza passare da gare. Come dico da sempre,

Mi riferisco, in particolare, al porto di Genova, per due semplici motivi. Come lei ben sa, il raddoppio del Canale di Suez ha creato delle condizioni estremamente particolari per il trasporto delle merci.

veicolare verso il nostro Paese fino a 700 treni al giorno (così è riportato nel progetto). Sappiamo che il Governo elvetico ha più volte cercato di stimolare il nostro Paese affinché Genova possa essere il terminale diretto di questa grandissima opera per il trasporto di merci su ferro.

Si può arrivare realmente a creare aree logistiche integrate che poi - si è fatto prima riferimento all'ultimo miglio - creano i presupposti per realizzare un'intermodalità.

dal 2007 in avanti. I tanti porti del nostro Paese, le poche opere (soprattutto nell'ultimo decennio), il problema delle autorizzazioni e delle manutenzioni straordinarie (si è fatto prima cenno ai fondali, ai dragaggi) e tutta una serie di questioni irrisolte rendono sempre meno competitivo il nostro sistema portuale. La mia domanda è relativa alla Puglia, che vive un problema di di sofferenza economica per le crisi delle aree industriali di Brindisi e Taranto. Il Governo come intende valorizzare le infrastrutture portuali esistenti, a fronte di opere che non sono state più realizzate in questi anni? Si pensi al dragaggio dei fondali del porto di Taranto,

con quali modalità vuole intervenire per valorizzare le infrastrutture portuali esistenti, sia le grandi che le piccole. Questo vale come micro esempio per la Puglia, ma può valere per tutta l'Italia.

ricordato sia il senatore Gibiino che il senatore Bruni; abbiamo un notevole problema di intermodalità e poi di corridoi, come ricordava il senatore Crosio. Dobbiamo perciò avere un approccio olistico al problema della portualità, considerandola un sistema economico, un sistema territoriale, un sistema di grandi potenzialità di crescita, perché oggettivamente le trasformazioni in atto, come il raddoppio del canale di Suez, danno

ci costano 40-50 miliardi, a seconda degli studi, ma il fatto di non coordinare, di non avere l'ultimo miglio ferroviario, di non coordinare i corridoi, di non renderli operativi, ci rende ovviamente un sistema debole.

Dobbiamo essere un sistema italiano diffuso, ma un unico sistema, certamente. Non abbiamo il grande porto su cui concentrarci, ma come sistema dobbiamo viverci e operare. Per questo abbiamo rafforzato nella riforma il ruolo di coordinamento centrale. Penso al porto di Taranto, una vicenda che ho seguito da vicino quando ero Sottosegretario e che ho continuato a seguire da Ministro. La crisi del porto di Taranto è dovuta al ritardo nell'esecuzione degli investimenti già autorizzati e finanziati; ritardi di dieci, dodici anni, in cui il terminalista poi scappa via. A

ma anche di approdo turistico, perché è un porto di grande potenzialità. Quindi, dobbiamo anche coordinare le funzioni e fare in modo che i porti siano multi funzioni e non mono funzioni, altrimenti rischiano molto in un mercato globale dove alcuni operatori determinano da soli

2015-2016, dove mettiamo a disposizione ulteriori 17 miliardi per lo sviluppo della rete ferroviaria, vi sono investimenti per quasi un miliardo per l'*upgrading* dei corridoi merci,

- attraverso il ferro *bonus*, l'altra misura di incentivo, di trasportare sempre più le merci dalla gomma al ferro. Spostare almeno il 30-40 per cento delle merci dalla gomma al ferro è un obiettivo strategico del Paese: vuole dire meno congestione, meno necessità di strade; vuol dire seguire la linea dei nostri amici e vicini, come gli svizzeri, per i quali il sistema dei tunnel rappresenta nelle nostre interlocuzioni un eccezionale sistema integrato con il porto di Genova.

le infrastrutture di ultimo miglio, l'R6 ha un programma di infrastrutturazione di ultimo miglio; penso ai lavori che stiamo facendo a Livorno, molto importanti, ma anche in altri porti, Taranto. Queste infrastrutturazioni dell'ultimo miglio sono il segno che pensiamo in termini integrati tra i vari sistemi: i porti non possono programmare i loro investimenti da soli,

promosso il *preclearing*, ossia lo sdoganamento in mare: più di 3.500 navi oggi vengono sdoganate direttamente in mare e ciò è stato molto apprezzato dagli operatori internazionali. Abbiamo 15 porti che ora fanno il *preclearing*, lo sdoganamento in mare.

Nord. Credo che il Paese sia in movimento, con i provvedimenti sui dragaggi, fatti insieme al Ministero dell'ambiente, con la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione in capo alle dogane, che hanno fatto uno straordinario lavoro, con la semplificazione della*governance*, con cui dai comitati portuali passiamo ai comitati di gestione. La senatrice Orrù pone un problema molto serio: non dobbiamo dimenticarci

- adottiamo anche, finalmente, un regolamento delle concessioni, che mancava da oltre dieci anni e che era necessario. Lo abbiamo predisposto, lo abbiamo mandato per le osservazioni ed è in fase di recepimento definitivo.

davvero abbiamo posto come uno degli elementi iniziali e più importanti, tant'è vero che siamo finalmente alla conclusione del dibattito sul regolamento delle concessioni e possiamo dedicarci a un sistema regolamentato dal centro in maniera adeguata. Ancora una volta, poiché ci diamo l'ambizione di avere comitati di gestione linea con le principali autorità portuali d'Europa, i criteri sono quelli di avere persone competenti, capaci, e che abbiano competenze manageriali. Non è necessario che abbiano che abbiano vissuto nel porto, ma è importante che abbiano competenze manageriali, perché il porto è anche una grande impresa. Ed è evidente che per noi le procedure di concertazione - si cerca ovviamente l'intesa con le Regioni su detta questione

un sistema che credo sia pronto. Speriamo di poter sviluppare questa economia del mare, così necessaria per promuovere l'occupazione e la crescita nel nostro Paese.

la richiesta che le abbiamo posto era ed è importante, proprio per garantire che ogni realtà territoriale possa davvero essere parte di questo sistema; un sistema che comunque noi immaginiamo già semplificato, perché la semplificazione Chiediamo però di valutare più attentamente questa tipologia di proposta, perché comunque i Comuni capoluogo hanno anche un'importanza territoriale un po' più vasta, oltre che per il Comune stesso che rappresentano. Quindi, chiediamo comunque di valutarlo come comitato, perché sarebbe realmente snello, ma per poter fare un lavoro di insieme e valutare tutto quello che è il sistema portuale,

non ci sono fondi pubblici da investire immediatamente, ma ci ha trasferito oggi la necessità di una consapevolezza, per cui cui la riforma della portualità deve essere accompagnata da una regia complessiva di tutto il sistema Paese. Ci rendiamo conto che un problema drammatico è quello dell'intermodalità e della connessione di ciò che giunge attraverso il mare nei porti (merce e passeggeri) e che deve essere poi trasferito

ha citato, perché tutto ciò funzioni; altrimenti perderemo competitività. Quel porto straordinario del Nord Europa di cui parliamo, Rotterdam, ha 96 chilometri di banchine, che sono correttamente collegate a un sistema

Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto di quanto ha detto, anche se purtroppo il *question time* ci obbliga a stringere temi complessissimi in tempi molto ridotti.

Non riusciamo inoltre a integrare i sistemi, che è il fatto fondamentale. Parlo ad esempio di Genova-Savona, che è assolutamente da fare nell'immediato, a mio giudizio.

Ministro, lei ha l'onestà di ammettere che dobbiamo rilanciare anche il sistema ferroviario, e questo deve essere un punto di partenza. In terzo

di questo importante sistema di trasporto ferroviario, che deve partire dal nostro Paese e ci sono le condizioni per lavorarci. Tiferemo per lei, mantenendo sempre il fiato sul collo.

se non c'è una politica economica di segno diverso, registreremo comunque un aumento del divario e una mancata diversificazione. Penso al traffico passeggeri, che al Sud potrebbe essere molto più florido. Pensiamo - ad esempio - agli itinerari delle navi da crociera, che prevalentemente utilizzano come scali di partenza e di arrivo quelli del Nord Italia, mentre il Sud viene usato*, en passant*, come meta turistica.